nell'esame del decreto-legge si coglie un pregiudizio che sfocia - inutile dirlo - nel reato di immigrazione clandestina, che, come abbiamo visto, verrà poi introdotto nel disegno di legge che esamineremo. Mi sembra chiaro che questo è l'orientamento del Governo, almeno fino qui: non si capirebbero, altrimenti, misure così drastiche, talvolta poco efficaci e, forse, inapplicabili, volte a lanciare messaggi sociali e politici, più che ad affrontare e risolvere alla radice i problemi. Ad esempio, le misure relative all'espulsione, che trasformano la violazione amministrativa in un reato penale, sono gravi, di difficile applicazione e possono rivelarsi dannose, perché contribuiranno a spingere fasce di immigrati irregolari verso la criminalità e ad intasare il lavoro della magistratura e delle carceri. Qualsiasi intervento di ordine penale, per altro, non si giustifica automaticamente per l'appartenenza ad una categoria, ma è relativo alla pericolosità del soggetto. Così, almeno, abbiamo cercato di sostenere nei nostri emendamenti, perché per tutti vige il principio per cui l'azione penale va accertata rispetto ad una persona che ha commesso il fatto, perché essa sia socialmente pericolosa (emendamento che abbiamo cercato di introdurre). Non vi può essere, perciò, la presunzione *ex lege* di una fattispecie predefinita di persona socialmente pericolosa, un prototipo. Questo travolge i principi dell'ordinamento penale e, sotto il profilo costituzionale, certamente è dubbio. Veniamo, poi, all'aggravante di pena, secondo la quale si introduce uno strano principio per cui il reato non è uguale per tutti, ma agisce in misura diversa per la condizione oggettiva di essere immigrato clandestino. Questo significa che la pena non è collegata alla tipologia del reato, ma della persona, per la condizione in cui essa viene a trovarsi. Certamente ci sembra un *vulnus* molto grave al complesso del nostro ordinamento. Non mi soffermerò su altri aspetti del decreto-legge che saranno trattati; voglio però precisare che ci siamo orientati in tutto il lavoro delle Commissioni - e lo rifaremo in Aula - con proposte di merito, senza alcuna pregiudiziale, volti a cogliere i fenomeni dell'insicurezza in vari campi, a non trascurare fatti che allarmano i cittadini, legati a reati commessi dagli immigrati, anche clandestini. Qui, però, occorre ristabilire un principio di realtà, più che una suggestione o un pregiudizio.

Questi sono i fatti che non sottovalutiamo, ma, alla luce di questi dati, è davvero fuorviante voler creare un binomio tra immigrazione e delinquenza, sbagliato politicamente, oltre che nella nostra funzione di legislatori. Abbiamo cercato, perciò, di immettere norme anche rigide, ma che evitassero, tuttavia, quelle qui previste. Abbiamo lavorato sull'articolo 5, per renderlo esigibile e concreto, non per trasformarlo in un incubo, nel caso si volesse affittare una casa ad un immigrato. La nostra intenzione è colpire lo sfruttamento e le situazioni illegali Pur tuttavia, su questo, come su altre norme (relative alla violenza sulle donne e sui minori), non è stata data una risposta convincente, perché alcuni fenomeni a noi sembrano allarmanti, in termini sociali e numerici, sicuramente anche di più di quelli che abbiamo trattato. Né si comprende perché vi sia stato il diniego su alcune misure antimafia che pure appaiono urgenti e necessarie. Ci preoccupa, però, soprattutto perché si è voluto rendere apparentemente più severo il provvedimento, ma, a nostro avviso, meno efficace, meno giusto e non proporzionale. Di fronte a fenomeni quali un'immigrazione così impetuosa, fenomeni europei e internazionali, molti si interrogano e cercano di trovare soluzioni. Purtuttavia, potremmo citare il caso della Spagna che ha aumentato del 45 per cento le espulsioni senza ricorrere all'aggravamento e al reato penale. Il fenomeno va affrontato, governato, ma in conformità con i princìpi costituzionali e le direttive europee. Rendere efficace il governo dei flussi, snellire la burocrazia della cosiddetta legge Bossi-Fini, che ha contribuito ad aumentare la clandestinità e il sommerso: poche, buone, efficaci norme, di questo avremmo bisogno e credo che lavoreremo per questo con severità, con serietà e complessità delle azioni anche qui in Aula, sperando di ottenere una legge giusta e buona per il nostro Paese.

*(PdL)*. Signora Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, lo Stato nazionale e il suo monopolio della forza sono le condizioni della democrazia, non sono un suo effetto, come avevano creduto nel loro stallo i colleghi nella precedente legislatura. La lotta contro la delinquenza, la delinquenza organizzata, la delinquenza sfusa, legata in qualche misura ai fenomeni dell'immigrazione, le connessioni tra l'una e l'altra e le loro contiguità politiche ed amministrative, è una lotta che si fa con lo Stato nazionale, con i suoi prefetti, quelli del conte di Cavour, di Spaventa, di Giolitti, colleghi della Lega; fa, colleghi della sinistra, con la retorica della società civile, di Hegel o di Gramsci che sia, della democrazia capace in quanto tale di risolvere con il suo solo dispiegarsi i temi della sicurezza o della lotta alla violenza. Proprio per quelli che erano stati su questo terreno gli inadempimenti, per non dire fallimenti, della precedente legislatura, il primo provvedimento di un certo respiro in questa legislatura, come è stato ben rilevato nelle relazioni di ieri, non poteva che investire questo terreno. Quando la scorsa settimana, colleghi della sinistra, l'onorevole Veltroni è venuto a Caserta e ha chiesto, in modo un po' metallico ma apprezzabile, che gli appalti nelle Province del Mezzogiorno fossero gestiti da comitati presieduti dai prefetti, ha riconosciuto che alla violenza e all'insicurezza della criminalità si può opporre solo la forza dello Stato, l'autorità dei prefetti del Risorgimento, e si trovava a Caserta. Non ha invocato bassolinismi, democraticismi di maniera le altre compagnie dialettali che hanno guidato la riforma costituzionale della XIII legislatura, quella fatta negli ultimi giorni a colpi di maggioranza, nella quale il termine Stato era l'ultima componente della Repubblica, dopo la Regione, gli enti locali e le Comunità montane. Ecco perché gli argomenti sviluppati ieri pomeriggio da alcuni colleghi sulla pregiudiziale di costituzionalità, mi sono sembrati, come ha detto con molta efficacia il senatore Longo, molto marginali, molto laterali, molto di maniera, molto comizieschi, tanto è vero che poi hanno dedicato gran parte del loro spazio alla questione delle televisioni di Berlusconi. Le questioni di costituzionalità sono questioni vere e serie e la nostra normativa, lo hanno rilevato molto bene i rappresentanti del Governo nel lavoro in Commissione, è legislazione di codice, quella legislazione alla quale, secondo Montesquieu - come si insegnava una volta -, ci si accosta con mano tremante e non più di una volta nel corso di una generazione, nel senso che ogni norma deve poi far sistema con un'altra, ogni termine, ogni riferimento con un altro termine e un altro riferimento. Da questo punto di vista le difficoltà che noi abbiamo incontrato erano proprio l'architettura dei criteri di necessità e di urgenza. Non tutti siamo soddisfatti, forse gli stessi rappresentanti del Governo, di come abbiamo sistemato le questioni sulle Commissioni. Personalmente mi auguravo che la *connection* con i problemi della sicurezza stradale in vista dell'estate, non per crociate di proibizionismo antialcolico ma proprio per i dati riferiti dalla polizia stradale, ricevessero *in re ipsa* carattere di necessità e di urgenza.

di aver affrontato problemi montesquieuiani di legislazioni di codice senza le opacità e, consentitemi di dire, le viltà che caratterizzarono il Parlamento nella scorsa legislatura.

e questo forse fa la differenza quando si parla di necessità e di urgenza e soprattutto di ciò che il popolo chiede a gran voce, così ci è stato detto sia nelle relazioni che in alcuni interventi da parte di Ebbene, questo Paese da quattro anni - e il Centro di ascolto radicale dell'informazione radiotelevisiva lo ha documentato - è bombardato da un'informazione drogata che più che raddoppiare, ha fatto triplicare, in alcuni casi, nelle reti Mediaset per l'appunto, ciò che ha a che fare con criminalità, cronaca giudiziaria e cronaca nera in prima serata, superando anche la politica che, sono d'accordo anch'io, dovrebbe porre al centro Montesquieu per quanto possibile. Purtroppo, invece, ci troviamo a doverci confrontare con questo stato di cose,

resta un Paese sostanzialmente sicuro. Quindi, voi avete voluto vendere, essendo il capo della vostra coalizione abituato a vendere sin da piccolo, un prodotto che nessuno voleva. Questo è modo avete dovuto cercare di limitare, aggravandoli, i problemi. Infatti, la criminogenità, cari colleghi della Lega, che ieri è stata tirata in ballo relativamente ad alcune politiche del Governo Prodi, è insita nella Bossi-Fini e nella Fini-Giovanardi. Quelle sono misure che creano crimine, non

dove esiste l'obbligatorietà dell'azione penale, nel giro di tre o quattro mesi tornerà ad essere ancora una volta il fanalino di coda in Europa per il rispetto dei diritti umani e ancora una volta in quell'emergenza giustizia

sullo Stretto di Messina e le centrali nucleari continueremo a invadere l'Italia di cemento perché solo così, da una parte, e con il diritto penale dall'altra, si possono arginare fenomeni che non siete capaci di governare. Questo è un Paese che avrebbe bisogno - e lo avete messo nel nome della vostra coalizione - di libertà e voi invece ci date lo sceriffo. Questo è quello che ci state proponendo, esclusivamente questo.

che su alcuni aspetti di questo decreto si sarebbe potuto fare meglio e si spera, grazie al dibattito parlamentare, di limitare i danni. Spero che il senatore Compagna si ricordi quel che ha detto quando si comincerà a votare. La speranza, almeno da questi banchi, è l'ultima a morire. Ieri sera eravamo pochi, come è stato fatto notare in conclusione di dibattito, e la senatrice Poli Bortone ha svolto un intervento di grande buonsenso politico e di grande umanità relativamente alla sua esperienza di amministratore in quanto sindaco. Invito i colleghi del PdL ad andare a rileggere tale intervento, perché è fondamentale recuperare tutto ciò che di positivo e quindi di velatamente critico esso conteneva, in quanto sicuramente la settimana prossima ci tornerà utile. Per quanto riguarda noi radicali, ci avvarremo della prerogativa di sindacato ispettivo perché i CPT rischiano di diventare tutt'altro, tutt'altro, dei veri e propri campi di filtraggio sul modello ceceno, se si dovesse portare a casa tutto ciò che avete inserito nel vostro pacchetto. Abbiamo creato un Intergruppo parlamentare di amicizia con i popoli rom e sistematicamente, dalla settimana prossima, inizieremo a visitare tanto i campi nomadi quanto i CPT, preparando anche proposte di legge per rimettere al centro i diritti di cittadinanza e non invece le armi nelle fondine dei vigili urbani.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, contrariamente all'esposizione del collega che mi ha preceduto, intendo sottolineare che il provvedimento in esame era lungamente atteso sia dai cittadini di questo Paese, sia dagli operatori della sicurezza e delle Forze di polizia. Da tempo e anche di recente, nel corso delle nostre audizioni parlamentari, lo stesso direttore generale della Pubblica sicurezza prefetto Antonio Manganelli ha posto in rilievo come l'operato meritorio di tutti i cinque Corpi di polizia dello Stato sia sostanzialmente vanificato da un reticolo di provvedimenti e leggi che tende più a giustificare chi commette reati che non a proteggere le persone oneste e operose che hanno reso grande la nostra Nazione. La gran parte dell'opinione pubblica del nostro Paese rifugge sicuramente dall'idea che si possa continuare con un politica del diritto a forte lettura ideologica, tesa più a perdonare i comportamenti devianti e criminali che non a prevenirli e reprimerli e, conseguentemente, a tutelare le vittime. Finalmente, con il provvedimento al nostro esame, riparte la stagione della tutela dei diritti, ma anche dei doveri. Legalità, diritti, solidarietà e Stato sociale sono i pilastri di una cultura occidentale dello Stato di diritto, che mette al centro del sistema giuridico di protezione la persona, i suoi diritti, i suoi bisogni. Ma alla parità dei diritti deve corrispondere la parità dei doveri tra tutti i soggetti che vivono in uno stesso territorio e in un medesimo ordinamento e fra questi diritti il rispetto della legge e l'adempimento degli imprescrittibili doveri di solidarietà riguardano sia i cittadini che gli stranieri. Lo scorso anno, caro senatore Perduca, sono stati denunciati in Italia 3 milioni di reati e conseguentemente sono state 3 milioni le vittime che hanno subito atti di criminalità. il titolo di questo decreto-legge, «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica», non costituisce solo una modifica semantica rispetto ad una politica legislativa che individuava questi provvedimenti come «misure urgenti a tutela dell'ordine pubblico», a tutela dell'ordine pubblico», bensì indica un mutamento di tendenza assolutamente importante e significativo. Non vi è libertà se non vi è sicurezza, e finalmente anche in Italia si afferma, con il decreto-legge in discussione, questa endiadi della tradizione costituzionale occidentale: libertà e sicurezza, i risvolti della stessa medaglia. Ricordo che sin dalla prima Carta costituzionale scritta, la *Magna Charta* del 1215,

La prima Costituzione scritta francese parla di libertà e sicurezza; di diritti di libertà e sicurezza parla il Trattato di Nizza ed il Trattato che adotta una Costituzione europea. Il diritto alla sicurezza quindi è un diritto a rilevanza costituzionale, che si traduce in un dovere dello Stato di contrastare con ogni strumento la barbarie della criminalità, che non è un prodotto indefettibile, ma solo il risultato dell'azione umana. Diritto alla sicurezza significa prevedere il ricorso a provvedimenti clemenziali solo quale *extrema ratio* e l'allarme sollevato dai vertici delle Forze di polizia deve essere preso con grande serietà, rifuggendo dalle tentazioni proposte in quest'Aula di ritornare alla stagione degli sconti, delle amnistie e degli indulti. Il perdono appartiene alla sfera etica degli individui, non all'azione laica dello Stato. Dobbiamo convincerci tutti che il reato è il frutto del disvalore sociale delle azioni delittuose individuali, non la conseguenza ineluttabile di una responsabilità collettiva o della società. Per la natura provvedimentale e d'urgenza di questo decreto-legge, che la Costituzione affida al Governo, non è questa la sede per affermare l'allargamento di ipotesi di reato dirette a contrastare nuove forme di devianza, contro le donne, i minori oppure per mitigare le conseguenze di nuove emergenze, ma è sicuro che con il disegno di legge collegato del Governo dovremo allargare la sfera di protezione di questi diritti. Deve essere chiaro che per questa maggioranza si impone in primo luogo la difesa di Abele e l'efficace tutela della *restitutio in integrum* alle vittime e non il contrario. Non si può rovesciare il sistema dei rapporti per proteggere Caino ed abbandonare Abele. È pur vero che la pena non potrà essere esclusivamente carceraria ma modulata secondo criteri moderni di meritevolezza e di efficacia, tuttavia l'efficacia della sua esecuzione rappresenta un elemento indefettibile della forza dello Stato affidata alla deterrenza penale e questi effetti dovremo riaffermare con i nostri provvedimenti. Se non vi è questa deterrenza non vi è diritto penale, che innanzi tutto è prevenzione con un'importante forza pedagogica. Signor Presidente, onorevoli colleghi, alcuni giorni fa in quest'Aula abbiamo rievocato il sequestro, l'omicidio e la strage dei poliziotti e dei carabinieri di scorta al presidente Aldo Moro. A distanza di trent'anni ho subito quasi una violenza psicologica nel ripensare a quei fatti tenendo conto che gli autori di quelle stragi, dopo qualche anno di detenzione carceraria, sono in libertà ed alcuni di loro sono persino stati assunti alle dipendenze dello Stato e della pubblica amministrazione. Dalla meritevolezza della pena siamo passati ai premi di Stato, ma non risulta che i figli dei colleghi poliziotti e carabinieri caduti nello svolgimento della loro professione siano stati assunti dallo Stato o dalla pubblica amministrazione: due pesi e due misure che segnano l'urgenza di cambiare radicalmente rotta. Deve essere chiaro a quei figuri, che non hanno mai risarcito, né le vittime, né lo Stato, né tampoco - molti di loro - hanno manifestato segni di resipiscenza, che il loro comportamento deve essere contrastato. Certo non penso alle persone che persino sono state elette ed elevate a questi scranni parlamentari; provo un po' di compassione per il loro comportamento. Credo però che per la maggioranza dei cittadini questi fatti non sono tollerabili, poiché costituiscono un grave difetto della nostra democrazia. La politica criminale non può essere gestita con quel perdonismo asseritamente dettato dalle esigenze di ordine pubblico negli istituti di pena, in relazione alla loro ricettività carceraria o ai benefici di chi è stato condannato. Le concessioni del sistema che riguarda i premi e soprattutto il trattamento penitenziario devono essere legate a princìpi di meritevolezza. In tutto questo scenario una riflessione si impone sul ruolo e sull'importanza che nel nostro Paese hanno avuto ed hanno le istituzioni spesso maggiormente colpite, come la magistratura e le forze dell'ordine. La morte l'altro giorno del sottotenente dei Carabinieri, rilevata dagli organi di stampa quasi come una fatalità, rende evidente questo *gap* culturale dei mezzi di comunicazione di massa in relazione al dovere di informare l'opinione pubblica. Stessa sorte ha avuto qualche giorno prima l'omicidio di un agente della Polizia stradale. Un piccolo spazio nella quotidianità giornalistica per grandi eroi, ma chi ripagherà mai le mogli ed i figli per l'amore e l'affetto immolati sull'altare della sicurezza dei cittadini? Signor Presidente, onorevoli colleghi, se si uccidono così facilmente gli appartenenti alle forze dell'ordine è anche perché il sistema penale appare oltremodo blando - per utilizzare un eufemismo - mentre l'arroganza e la soverchieria della criminalità sono sempre più evidenti e per questo non possiamo arrenderci all'idea che siano fenomeni incontrastabili e incontrollabili. C'è davvero bisogno di domandarsi quale pena in astratto potrà essere irrogata agli autori dell'omicidio del nostro ufficiale dei Carabinieri e se le norme oggi in vigore sono davvero efficaci. La risposta fornita dall'ordinamento è quasi pleonastica. Con qualche anno di reclusione, tra giudizio abbreviato, patteggiamento in appello,

che se non si riuscirà a riaffermare l'idea che lo Stato di diritto prevale sulla criminalità in ogni sua forma non si riuscirà neanche a riavviare il nostro Paese verso i suoi più alti ed immancabili destini. Questa è

dei provvedimenti normativi inseriti nel decreto-legge in conversione essendo gli stessi la ripetizione, anche nelle virgole, delle analoghe norme contenute nei disegni di legge nn. 582, 583 e 617,

aprire il dibattito e quindi accogliere gli emendamenti da noi proposti in materie quali il maltrattamento contro familiari e conviventi, l'adescamento dei minorenni attraverso la rete Internet, il delitto di impiego di minori nell'accattonaggio, gli atti persecutori, l'aggravante del reato di truffa in danno di soggetti deboli come nel caso degli anziani, il vandalismo nei centri urbani, subordinando la concessione del beneficio della sospensione della pena all'eliminazione dei danni, l'aumento del potere dei sindaci in materia di occupazione di suolo pubblico al fine di commercio abusivo, l'aggravamento dei reati di discriminazione e violenza per motivi di odio razziale, religioso e omofobico. Nessuna di queste nostre proposte, come delle ulteriori proposte da noi condivise presentate dal Partito Democratico, è stata presa in considerazione.

a fronte della negazione di apertura di discorso, di confronto, di introduzione di norme su fenomeni criminali crescenti, di cui i cittadini soffrono e su cui era necessario ed urgente intervenire, il Governo e la maggioranza hanno invece ritenuto importante ed urgente, anzi urgentissimo, introdurre il cambiamento del nome dei centri di permanenza temporanea. Il termometro della sensibilità sui temi che interessano i cittadini è proprio in questo; noi insisteremo in quest'Aula perché vengano prese in considerazione le nostre proposte, ritenendo insultante per il Paese che si ritenga urgente cambiare il nome dei centri e non intervenire

necessità di addivenire ad un provvedimento che risponda alla domanda di sicurezza ci sia una larghissima condivisione. Mi pare che i lavori di Commissione abbiano dimostrato una grande partecipazione anche dell'opposizione

ma le intenzioni c'erano. Il Paese sta chiedendo maggiore tranquillità, i cittadini pretendono un certo rispetto per il loro modo di agire ed il loro modo di relazionarsi, e pretendono un po' più di sicurezza. Come Lega Nord, centrodestra, PdL, ci siamo impegnati di fronte al nostro elettorato, di fronte agli italiani e questo è il nostro modo di onorare gli impegni, uno dei primi provvedimenti che si affrontano è proprio per dare risposta ai loro bisogni. Senza approfondire ogni aspetto, mi fermerò su un punto che mi sta particolarmente a cuore: siamo contenti

quasi tutto può fare un'amministrazione comunale: può accedere a tutte le banche dati di questo Paese, può sapere di tutto su qualsiasi cittadino di qualsiasi Comune italiano, può conoscere la sua situazione patrimoniale e la ultima dichiarazione dei redditi, ma non può sapere, per esempio, se è stato condannato, se è in procinto di esserlo, cioè la situazione che più interessa perché magari i vigili municipali possano cooperare col sistema delle forze dell'ordine. Altra cosa che ci è stata chiesta è la certezza della pena, perché in questo Paese sembra che i codici penali esistano, siano scritti, ma poi siano sistematicamente ovviati*,* ovviati*,* bypassati, sospesi, dalla legge Gozzini in poi. Noi conosciamo il nostro sistema e il nostro ordinamento. Da quando nacque si pose una grande dicotomia: che tipo di strada intraprendere? Quale funzione dovrà avere la pena? Le grandi correnti erano la retribuzione o la rieducazione: tanto male fai, tanto male dovrai avere, oppure tentiamo di recuperare anche chi sbaglia. Ebbene, il nostro Paese

Premesso questo, vengo ad un punto che al sottoscritto sembra abbastanza importante. È difficile

guidando un autoveicolo in condizioni di non poterlo guidare, sotto effetto dell'alcool (e fermiamoci all'alcool) e chi

Se si volesse trasformare tale pena, considerando la tenuità del fatto e il non aver commesso assolutamente niente di socialmente pericoloso, a noi sembrerebbe una cosa fattibile. Presenteremo degli emendamenti in Aula in tal senso e preghiamo l'Aula, ma anche il Governo, di essere attenti su questa tematica.

onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo (anche se ne vedo pochi oggi), l'irregolarità e la clandestinità non sono sempre frutto di una scelta consapevole dell'immigrato. In molti casi sono il combinato di una condizione sociale e di lavoro, lavoro in nero e lavoro sommerso, dovuta alle conseguenze di un bisogno per chi intraprende il cammino della speranza e dovuta alle conseguenze di uno sviluppo distorto che è tutto nostro. Dovuta in particolare ad una legge sugli ingressi e il soggiorno nel nostro Paese, la famosa legge Bossi‑Fini, carente e inadeguata alle esigenze attuali. Vorrei perciò riflettere con voi sul fatto che, nel momento stesso in cui parlate di tolleranza zero nei confronti degli immigrati irregolari clandestini, pensare anche ad aggredire con forza il fenomeno del lavoro nero e del lavoro sommerso, che sono sempre temi di alto allarme sociale nel nostro Paese. A questo riguardo credo che non ci possono essere due pesi e due misure. e due misure. Quando viene scoperto questo grave sfruttamento scattano i provvedimenti di sanzione per l'imprenditore o per l'intermediario di manodopera che si è macchiato di un reato, ma la vittima viene equiparata al criminale, viene privata della sua libertà e scatta automaticamente il provvedimento di espulsione. Dopo il danno, il grave sfruttamento e lo schiavismo, la beffa della detenzione e del rimpatrio, che tra l'altro si vuole estendere anche alle prostitute. Agendo in questo modo, vedete, voi ci proponete un sistema sociale e giuridico retto dalla legge del più forte. Un sistema che alla lunga può essere molto rischioso e pesante da sostenere anche per il più forte. Si tratta, infatti, di un'operazione rischiosa perché accentua le disuguaglianze e aumenta l'incomprensione tra italiani ed immigrati, configurando per il nostro Paese (che ha una sua peculiarità rispetto a tutti gli altri) una sorta di politica immigratoria *à la carte*, una specie di politica del tipo usa e getta. La misura di espulsione anche per noi è legittima all'interno di uno Stato di diritto, ma è altrettanto vero che va inquadrata in un contesto che non prefiguri le espulsioni di massa che si stanno prefigurando per il nostro Paese. Siamo in presenza di misure per certi aspetti insensate: insensate perché l'espulsione non è più un fatto unilaterale, fatto unilaterale, ma coinvolge più parti, più Paesi e perciò il dialogo e la cooperazione con i Paesi di origine e di transito sono strettamente interconnessi. Senza questa cooperazione - badate - non c'è espulsione che tenga. Mi chiedo e vi chiedo, allora: cosa succede all'immigrato tenuto nei centri di detenzione se non arriva il nullaosta dal Paese di provenienza? Dopo 18 mesi dovrete anche liberarlo. Urge quindi la necessità di stabilire accordi complessivi con i Paesi di provenienza per ottenere una effettiva cooperazione in materia e per rendere più efficace l'istituto delle espulsioni. Il punto vero del vostro pacchetto sicurezza in materia di immigrazione è quello di anteporre interessi di parte ad un problema di gestione reale. Le vostre risposte mirano alla riduzione degli spazi di libertà e giustizia non solo per gli immigrati, gli zingari e le prostitute, ma anche per i cittadini comunitari. L'automatismo, infatti, tra condanna e provvedimento di espulsione che volete introdurre anche per i cittadini comunitari ha questo fine. Il fatto che le vostre proposte in materia di espulsione di cittadini di Paesi terzi non tengano nel dovuto conto, così come fanno gli altri Paesi europei, elementi quali la durata del soggiorno dell'interessato e i suoi legami con il Paese di origine ne è un'altra prova. Ancora, la riduzione dell'ambito di applicazione del ricongiungimento familiare che proponete nell'apposita proposta di decreto, oltre ad essere lesiva dei principi comunitari di non discriminazione costituisce un freno al processo di integrazione. Il nostro Paese, a questo punto, ha bisogno di integrazione, proprio per assicurare sicurezza e legalità non solo agli italiani, ma anche agli immigrati. *(Applausi

Fra questi certamente c'è il diritto alla vita, che implica il diritto alla sicurezza nella propria abitazione, nella propria vita quotidiana e nel proprio lavoro.

un'invenzione dei media, come qualcuno ha detto, non è un allarme ingiustificato: basta parlare con i cittadini della loro vita quotidiana, basta analizzare i dati sui reati, basta pensare anche alle spese che molti cittadini affrontano nel tentativo, spesso vano, di garantire la propria sicurezza. Ecco perché è fondamentale aver iniziato con questo difficile tema. È un tema difficile, tant'è vero che i provvedimenti che si intendono porre in atto sono stati suddivisi in un decreto-legge

anche in un tema come questo, mantenere le caratteristiche che deve avere un decreto-legge. Non si può inserire nel decreto-legge tutto ciò che si ritiene positivo, ma deve essere, per l'appunto, necessario ed urgente.

espressione di un Governo ‑ quello che vi era in Italia quattro secoli fa - che, non riuscendo ad arginare realmente il crimine, reprimeva in modo arbitrario e generico cose che crimine non erano.

la verità in tasca.

animerà il lavoro dell'Aula: quanto più questo avverrà, tanto maggiori saranno gli effetti positivi che tutti ci proponiamo dal provvedimento al nostro esame.

una nuova finestra"). L'ordine del giorno reca: «Informativa urgente del Governo sui recenti fatti accaduti presso la clinica Santa Rita di Milano». Dopo l'intervento del rappresentante del Governo, ciascun Gruppo avrà a disposizione cinque minuti.

Santa Rita è una casa di cura privata, accreditata e a contratto, dispone di 276 posti letto di degenza, di un dipartimento di emergenza e accettazione, di circa 700 dipendenti e di un poliambulatorio con molteplici specialità mediche e chirurgiche. Le risorse assegnate alla casa di cura Santa Rita nel 2007 ammontano a 42 milioni di euro per i ricoveri e a 11.181.000 per l'ambulatoriale. La casa di cura Santa Rita è stata oggetto, a partire dal 1999, di un progetto di ampliamento strutturale, che ha comportato negli anni un significativo incremento di posti letto disponibili nella struttura (dai 38 del 1999 agli attuali 276). Passiamo ora a considerare gli avvenimenti che hanno riguardato la casa di cura Santa Rita nel 2007. Nel corso del 2007 sono state avviate dalla magistratura indagini sull'attività sanitaria presso la casa di cura Santa Rita che si riferiscono prevalentemente a fatti verificatisi negli anni 2005-2006. La Regione Lombardia e la ASL, nell'ambito dei rapporti instauratisi da tempo, hanno subito fornito la disponibilità a collaborare per quanto di loro competenza con la magistratura. A seguito di controlli effettuati dalla ASL città di Milano, questa ha inviato, in data 25 settembre 2007, alla procura della Repubblica gli esiti della relazione dei propri esperti e il giorno successivo è stata sospesa l'autorizzazione per l'attività di chirurgia toracica, dovuta alla mancanza di adeguati protocolli clinico operativi del quartiere operatorio, in particolare per quanto riguarda la gestione dei pazienti con infezioni acute in atto. in atto. Dopo gli interventi effettuati nella struttura e le ulteriori verifiche ad opera della ASL, nel mese di dicembre è stata revocata la sospensione dell'autorizzazione. Peraltro, nel corso del 2007, le verifiche del nucleo operativo di controllo della ASL hanno portato ad una rettifica della valorizzazione delle prestazioni di ricovero, non riconoscendo come rimborsabili prestazioni per circa 1.200.000 euro. Inoltre occorre ricordare che la legge attualmente in vigore, che è riferibile alla finanziaria 2001, prevede un controllo analitico annuo di almeno il 2 per cento delle cartelle cliniche, a fronte del quale la Regione Lombardia ha attualmente in essere operazioni di controllo per circa il 5 per cento delle cartelle cliniche. Vediamo ora le azioni attivate a seguito degli attuali avvenimenti. La ASL di Milano ha sospeso immediatamente il contratto di servizio in considerazione del fatto che i reati, in quanto di significativa gravità, sono stati contestati non solo alle persone fisiche ma anche alla persona giuridica. In esecuzione del sequestro cautelare disposto dal provvedimento giudiziario, la ASL ha inoltre provveduto a sospendere il pagamento delle prestazioni fino ad un importo pari al 50 per cento in più dalle somme oggetto di sequestro.

276 posti letto, un poliambulatorio e un dipartimento di emergenza e accettazione nell'area milanese, che impegnano la Regione Lombardia affinché siano soddisfatte le richieste dei cittadini interessati, in modo tale che i disagi per gli stessi siano ridotti al minimo. riguarda le azioni attivate dal Ministero del welfare, abbiamo innanzi tutto inviato due funzionari in veste ispettiva per collaborare alle verifiche messe in campo dalla Regione Lombardia, i quali ci riferiranno probabilmente nel corso della giornata odierna. Onorevoli senatori, è chiaro ed evidente che il Governo non ritiene di avere risolto il problema mandando un ispettore. Il punto non è chiudere la stalla dopo che i buoi sono scappati, ma bisogna evitare che questi episodi si ripetano in futuro. In particolare i fatti di Milano aprono una serie di interrogativi inquietanti:

sede, non è questo certamente il momento per discutere a fondo tutti i problemi sollevati, che però sono all'attenzione del Governo e che il Governo è disponibile a discutere nel dettaglio in qualsiasi momento e nelle opportune sedi referenti. Mi sembra giusto, però, affrontare brevemente alcuni di questi aspetti anche per dare un'indicazione di come il Governo intende muoversi al riguardo nel prossimo futuro. Anzitutto, il Ministero intende procedere in tempi brevissimi

affiancare ai controlli campionari il controllo sistematico su tutte le cartelle cliniche relative alle prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza, rispetto sia ai medici prescrittori che alle strutture erogatrici (e abbiamo gli strumenti per identificare queste prestazioni). Soprattutto, credo sia importante vedere quali azioni di sistema il Governo intende intraprendere; di costruire di concerto tra Stato e Regioni un sistema di qualità in sanità che preveda un controllo delle singole prestazioni e non solo la valutazione di standard.

opportuno creare in particolare un sistema informatizzato che consenta in tempo reale a Regioni e Ministero il controllo e la valutazione sistematica di parametri quali il rischio clinico, le procedure diagnostiche e terapeutiche con particolare riferimento alla qualità delle stesse, le risorse, le tecnologie, la *customer satisfaction* e quant'altro possa essere ritenuto utile. A questo proposito abbiamo insediato un gruppo di lavoro ristretto e informale (cinque persone estremamente qualificate) che già da tre settimane, quindi ben prima che emergesse il problema, sta lavorando ad un piano per implementare al più presto un sistema di informatizzazione per il controllo e la gestione delle procedure sanitarie in tutto il territorio nazionale. Questo gruppo sta già elaborando un progetto specifico per i sistemi di CUP (Centro unico di prenotazione) per abbattere le liste di attesa, l'introduzione di un fascicolo sanitario elettronico multidimensionale che rappresenti il percorso del paziente e non sia quindi una mera raccolta di dati e infine metodologie di telemedicina. Un altro degli aspetti già esistenti nel programma di Governo è la revisione dei criteri di accreditamento e selezione degli erogatori. Stiamo prevedendo come prime e immediate misure, legate anche all'abbattimento delle liste di attesa, la creazione di un accreditamento ulteriore, una specie di «bollino d'oro», con criteri molto più stringenti (ci si riferisce all'*assessment* tecnologico, ai controlli di qualità, alle dimensioni dell'attività clinica di eliminare la microsanità, che sappiamo essere quella meno virtuosa) da introdurre subito e che dovrebbe progressivamente - questa è l'idea - sostituire gli accreditamenti precedenti con un programma da concordare con le Regioni. Infine, un'altra considerazione emergente dalle vicende della casa di cura Santa Rita è quella della trasparenza e della pronta disponibilità di informazioni dettagliate ai pazienti relative alle indagini cliniche e strumentali effettuate e alle terapie messe in atto, in ogni momento del loro percorso nella struttura sanitaria. sanitaria. Quindi, i pazienti devono poter richiedere ed avere subito giudizi diagnostici, cartelle cliniche, esami strumentali, radiografie di laboratorio, preparati istologici e quant'altro. Questo aspetto, particolarmente importante ai fini della trasparenza delle prestazioni e di un reale controllo, potrebbe essere oggetto di appositi provvedimenti attualmente allo studio di questo Ministero.

pubblico e anche di tanti anni di lavoro come assessore regionale alla sanità della Valle d'Aosta. Siamo sicuri che la magistratura accerterà con precisione l'accaduto e che certi toni saranno smorzati perché credo, come medico, al senso di responsabilità

Pur essendo favorevole al privato in sanità come termine di riferimento per il funzionamento delle strutture pubbliche, ritengo che dobbiamo considerare l'esigenza di modificare i sistemi di accreditamento delle strutture private e porre in atto meccanismi di controllo della qualità dei servizi effettuati.

l'accreditamento dato dalla Regione in cui la struttura sanitaria privata si situa non può valere anche per tutte le Regioni vicine, che hanno una programmazione sanitaria differente.

intanto, l'appropriatezza delle pratiche, eseguite secondo linee guida ben definite; non può esistere un sistema di pagamento a prestazione effettuata; effettuata; l'accreditamento di una struttura privata non può prescindere dalla presenza nella stessa di alcuni servizi necessari alla completezza del percorso di cura, cosa che non avviene in tutte le strutture private accreditate. Il privato convenzionato non può infatti scegliersi - e in molti casi è così - solo alcuni settori di intervento, lasciando le patologie più gravi a carico del pubblico; non può indirizzare la sua attività su un *target* di pazienti e indirizzare i cronici, gli anziani, i diabetici, i malati acuti da pronto soccorso, le complicanze chirurgiche a carico del sistema sanitario nazionale: signori Sottosegretari, ciò non avviene in tutti i privati convenzionati, ma in molti in molti sì. Chiediamo quindi di modificare le regole di accreditamento delle strutture private e di fissare in modo preciso linee guida per le singole patologie, in modo tale che queste non siano dettate solo da esigenze economiche. Da questa revisione dei meccanismi attuativi deriverà sicuramente, a nostro parere, un miglioramento della qualità delle prestazioni offerte sia dal servizio privato che da quello pubblico.

Ci aspettavamo un giudizio di ordine generale anche sulla sanità italiana e su come cercare di tamponare questi malcostumi che non sono solo di Milano. Permetteteci almeno, colleghi, di interpretare l'indignazione e la rabbia della gente di fronte a certe notizie e la vicinanza alle famiglie di chi è stato utilizzato e strumentalizzato per un'opera prettamente mercantile, di fronte a questa che

Non vogliamo fare nessuna strumentalizzazione, signor Sottosegretario, lo dico con estrema lealtà, perché ci sono casi dall'una e dall'altraparte, al Nord e al Sud, ma vogliamo svolgere una seria riflessione.

Certo, 102 miliardi di euro fanno gola a tutti. Tutti però ci dimentichiamo del cittadino debole: un cittadino, quando entra nel tunnel della malattia, come diceva un ex Ministro, diviene il più debole. Dovremo essere - noi lo siamo tutti dalla parte del cittadino e lotteremo fino in fondo. Ecco perché, signor Sottosegretario, credo che la corsa ai DRG, il mercatismo, come lo chiama qualcuno, nella sanità vada

Presidente, egregi rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, è fuori discussione che la vicenda di cui stiamo dibattendo oggi rappresenti una pagina oscura e vergognosa della nostra sanità, ma ancor più un episodio umanamente, eticamente e civilmente deprecabile. Esprimo, a titolo personale ed a nome del Gruppo della Lega Nord, il più assoluto disprezzo nei confronti degli autori di simili nefandezze, che dimostrano che quando la salute viene interpretata a fini di lucro da parte di individui senza scrupoli, ogni delitto risulta possibile e l'animo umano riesce ad esprimere atti di sciacallaggio addirittura inimmaginabili. A tale proposito esprimiamo alla magistratura ed all'ASL di Milano, che sta fattivamente collaborando con essa, la più fervida richiesta di far luce su questo e su tutti gli episodi che possano essere ricondotti ad atti di tale sciagurata interpretazione sanitaria, affinché possano essere estirpate tutte le mele marce, che rischiano di screditare un sistema sanitario di rara efficienza come quello lombardo, esempio di assoluta eccellenza a livello europeo e mondiale, ove si coniugano mirabilmente professionalità, qualità e corretta gestione delle risorse, con efficacia ed appropriatezza. La dimostrazione della bontà di questo sistema non è riferibile ad una sensazione, ma risulta scientificamente da dati incontrovertibili, che vedono la Regione Lombardia erogare circa 14 milioni di prestazioni annue su una popolazione di circa 9 milioni. Pur ammettendo un'improbabile prestazione annua per ogni cittadino lombardo, risulta evidente che almeno 5 milioni di prestazioni vengono erogate a beneficio di pazienti provenienti da altre Regioni,

rimborsati solo parzialmente e con considerevoli ritardi, spesso di anni. L'assessorato alla sanità della Regione Lombardia, unitamente all'ASL di Milano, già nel corso dello scorso anno aveva intensificato i controlli procedurali e sui protocolli operativi nei confronti della casa di cura Santa Rita e di altre 4 strutture, alla luce di dati sospetti che avevano indotto ad una sospensione dell'autorizzazione all'esercizio

saliti alla ribalta della cronaca, ritengo tuttavia doveroso lanciare un monito affinché la situazione non subisca strumentalizzazioni e le colpe non vengano generalizzate; soprattutto evitare che un fatto isolato o eventuali successivi episodi estemporanei di malcostume e delinquenza creino allarmismo e vadano ad inficiare la fiducia del cittadino nella nostra sanità, che rimane comunque di elevata qualità. Ancor più rilevante è la serenità di non sentirsi *sub iudice* da parte di quelle decine di migliaia di operatori sanitari, dai medici agli infermieri, a tutte le figure sanitarie che con estrema professionalità ed assoluta dedizione continuano quotidianamente, tra mille difficoltà normative e strutturali, a garantirci il bene supremo della salute.

Fazio, mi dichiaro molto insoddisfatta perché mi sembra che dalle sue parole non emerga innanzitutto il grave allarme che questi fatti hanno determinato nell'opinione pubblica, per la crudeltà e il cinismo che hanno messo in evidenza e non certo per le strumentalizzazioni che

Quindi, né la clinica, né la Regione Lombardia possono essere considerate degli osservatori esterni. È una vicenda che si snoda nel tempo e che aveva dato ripetutamente segnali di irregolarità che avrebbero dovuto essere raccolti. Per ammissione dello stesso direttore generale dell'assessorato alla sanità regionale, già nel 2003 il notaio Pipitone, proprietario unico e legale rappresentante della clinica in questione, era ricorso al TAR contro la Regione Lombardia per avere il premio che era stato istituito a titolo di riconoscimento per le strutture ospedaliere la qual cosa crea in noi un certo stupore, perché viene spontaneo chiedersi perché premiare chi fa solo il suo dovere, cioè rispettare le regole. In quel medesimo periodo i cittadini della zona mettevano in atto una protesta molto forte, che io allora come consigliere regionale ricordo di aver raccolto, contro la decisione del Comune di Milano e della regione Lombardia di consentire l'ampliamento della struttura ospedaliera. Infatti lei, Sottosegretario, ha parlato di questa piccola clinica con 33 posti che è diventata di 220 in una zona congestionata, priva di infrastrutture viarie, priva di parcheggio e già congestionata da altre strutture ospedaliere. Inoltre, una domanda che sorge spontanea è come sia possibile che, mentre la magistratura indaga su fatti avvenuti tra il 2005 e il 2006, in quel periodo la ASL di Milano non abbia riscontrato alcuna anomalia, se è vero, come oggi riferiscono i giornali, che i morti al Santa Rita sono stati nel 2006 circa 336 e che in base all'età media dei ricoverati questa clinica ha il numero più elevato di morti. Purtroppo, solo nel 2007 la regione Lombardia interviene sospendendo l'accreditamento per la chirurgia toracica ed in seguito il primario del reparto viene sostituito. Sottolineo, allora, che vi è un'eccessiva proliferazione di strutture specialistiche ad alto livello in Lombardia: basta pensare che le cardiochirurgie assommano a 23, quando l'Inghilterra ne ha nove e questo favorisce la caccia al malato e abbassa il livello di appropriatezza e di sicurezza. La Regione è stata interessata da un numero considerevole di fatti gravi di truffa ai danni della pubblica amministrazione e anche con conseguenze gravissime per le persone malate: mi basta ricordare il caso Poggi Longostrevi (ho anche fatto parte della commissione d'inchiesta regionale ad esso dedicata) il caso Galeazzi, in cui morirono 11 persone perché la camera iperbarica veniva usata come un pullman, perché rendeva molto, e molti altri casi, di cui l'ultimo è la vicenda del San Raffaele. Inoltre, il comandante delle Fiamme gialle, Cesare Marangoni, dichiara che ci sono altre quattro strutture nel mirino degli inquirenti. Per questo il presidente Formigoni non può solo dichiararsi parte lesa, ma deve assumersi le sue responsabilità per quanto accaduto. Qui non si tratta di casi fisiologici per un sistema perfetto: qui c'è una patologia diffusa, che quantomeno ci interroga su quali sono gli obiettivi del sistema sanitario lombardo, se prevalga l'aspetto unicamente economico o se prevalga il diritto costituzionale alla salute. Occorre domandarsi come mai le ASL, dedicate unicamente all'acquisto dei servizi, alla programmazione e al controllo, non siano nelle condizioni di esercitare un controllo reale sulle strutture sanitarie perché sia consentito il pendolarismo, quando viene di fatto messo un tetto alle prestazioni a livello regionale e non altrettanto avviene per quelle a beneficio dei malati che provengono da altre Regioni:

non si preoccupa per le liste d'attesa che si allungano, perché ci sono tanti cavalli in regione Lombardia e poca erba, quindi l'erba bisogna prenderla da altre Regioni. senza nulla togliere all'eccellenza del sistema sanitario lombardo, che è storico, dato che da alcuni decenni in questa Regione si sono sviluppati centri pubblici e privati di rilevanza nazionale,

non sono contro i DRG, dico solo che vanno rivisitati perché alcune anomalie, come l'aumento del 104 per cento delle artografie in un anno in Lombardia va assolutamente rivisto (parlo della Lombardia perché è la realtà che conosco meglio). PRESIDENTE. Senatrice

con una messa a confronto dei diversi criteri di accreditamento che ci sono in ciascuna Regione. Infine, lei ha parlato di come viene attuata l'informazione dei cittadini, ebbene le confermo, anche per esperienza personale, che il consenso informato è un atto unicamente burocratico,

voglio innanzitutto ringraziare il sottosegretario Fazio per l'esauriente, puntuale e soddisfacente relazione sui gravissimi e inqualificabili avvenimenti nel caso della clinica Santa Rita di Milano.

XV legislatura, attraverso attività istruttorie, relazioni del nucleo investigativo, audizioni dei magistrati, dell'assessore regionale alla sanità della Lombardia e del direttore generale, con i quali abbiamo intrattenuto stretti rapporti fino all'interruzione della legislatura. materiale acquisito risulta, per decisione congiunta della Commissione e dei magistrati, secretato agli atti. Tuttavia, non violiamo nessun segreto ribadendo che è stata proprio l'azione di controllo della Regione, tra le poche in Italia ad eseguire controlli routinari ben al di sopra di quanto previsto dalle leggi, a sollecitare l'iniziativa giudiziaria e tutto quanto ne è scaturito. Va subito aggiunto che dalla Regione fu allora, contestualmente, sospeso l'accredito per quel reparto e sospesi i sanitari implicati. Le gravi violazioni erano abbastanza evidenti controllando l'appropriatezza degli interventi e delle cartelle cliniche. Le intercettazioni avranno fornito ulteriori certezze, se i provvedimenti restrittivi sono scattati solo ora; ma se pare abbastanza evidente, pur nel rispetto delle garanzie dovute, la grave responsabilità criminosa dei sanitari implicati non mi pare altrettanto evidente la responsabilità oggettiva della clinica, per la quale sarà importante attendere con rispetto le determinazioni dei gradi di giudizio. Ciò detto, non è possibile accettare la strumentalizzazione e la demagogia, che vedrebbe la Regione Lombardia, tra le più virtuose nei controlli, nei conti economici, nel rispetto delle liste di attesa, nell'emergenza-urgenza e in tutto quanto attiene anche al sistema sociale, additata tra i responsabili. Ancor meno accettabile è l'allarmismo che si vuol suscitare sul servizio sanitario nazionale, che tuttora l'Organizzazione mondiale della sanità definisce tra i migliori al mondo, da cui passano ogni anno nove milioni di cittadini e che pone la nostra Nazione tra quelle con maggior aspettativa di vita al mondo. Ancora meno accettabile è la disputa tra pubblico e privato.

l'azione di grandi istituti privati, quali il San Raffaele di Milano, che abbiamo luoghi di cura all'avanguardia. Il settore privato investe, rischia in proprio

Noi ringraziamo il sottosegretario Fazio per i provvedimenti proposti sui controlli e auspichiamo un'agenzia veramente terza, che regoli la domanda, che calmieri l'offerta, che controlli la trasparenza delle nomine e prevenga le situazioni di rischio. Concludendo, noi rifiutiamo le interpretazioni errate dell'articolo 32 della nostra Costituzione. non prevede uno Stato padrone che stabilisce dove i cittadini devono essere curati, da quali medici e di quali malattie devono ammalarsi; esso non prevede che lo Stato sia l'unico erogatore, organizzatore, produttore e controllore della salute. La nostra Costituzione prevede, invece, che lo Stato garantisca le regole, i requisiti, il riequilibrio delle diverse fortune delle Regioni ed i controlli garantiti. Nell'ambito di queste, tutti gli erogatori devono avere l'opportunità di offrire i propri servizi, tra i quali il cittadino deve essere rimesso al centro del sistema per poter esercitare il proprio diritto e la propria libera scelta. *(Applausi dal